concessioni per sei anni, con un rinnovo di altri sei. Era un risultato soddisfacente, e comunque importante. Ora, di fronte all'avvio di una

Non ci sono nei nostri concorrenti - Grecia, Spagna, Francia, ovvero i principali *competitor* del nostro sistema turistico - realtà come la nostra;

Credo che gli stabilimenti balneari rappresentino qualcosa di più di questi comparti; senza nulla togliere a questi ultimi, sicuramente per l'Italia rappresentano un qualcosa in più. Se il Governo va in Europa con il supporto di tutto il Parlamento,

europeo. Sul nostro demanio marittimo c'è un'ampia diffusione di stabilimenti balneari che sono diversi per specificità e per servizi da Nord a Sud, perché l'Italia è lunga e perché la concezione del turismo deve ancora decollare in alcuni ambienti e in alcuni settori, e quindi le imprese si caratterizzano con modalità diverse.

e soprattutto la salvaguardia del mare e delle coste, che spesso sono minacciate non solo dall'erosione ma, in questi ultimi tempi, anche da atti di vandalismo, nei confronti dei quali gli stabilimenti balneari sono un vero e proprio presidio in quanto tutelano anche il bene paesaggistico ambientale, in questo caso la spiaggia, la costa e il mare. e il mare. Questi stabilimenti svolgono dunque una finalità pubblica (sicurezza a mare, pubblica incolumità, salvaguardia del profilo costiero e paesaggistico, tutela dell'ambiente), quindi costituiscono un modello turistico che ha una sua tipicità che va salvaguardata. salvaguardata. Nel tempo abbiamo avuto una serie di leggi che si sono incrostate l'una sull'altra senza fare definitivamente chiarezza, fino alla direttiva europea Bolkestein,

una volta data la concessione con criteri per i quali si prevede una preferenza, c'è poi il diritto di insistenza. Quindi la concessione non è vita natural durante ma quasi, consentendo agli operatori di fare degli investimenti produttivi e di qualità in questi stabilimenti che offrono servizi di alta specializzazione di *comfort* e tutela, che fanno della nostre spiagge e del nostro settore turistico uno dei settori trainanti della nostra economia.

impone al Governo italiano una seria riflessione sulla situazione che di fatto si sta determinando. Infatti, per quanto riguarda le concessioni a scadenza, che queste vengano assegnate con gara, e quindi non siano più destinate a chi le aveva prima, comporta una situazione di scarsissima tranquillità degli operatori

di uscire dalle norme strette della direttiva Bolkestein - come è stato fatto per altri settori - per procedere successivamente ad una normativa quadro che regoli la materia, che da tempo immemorabile è oggetto di contestazioni,

per gli investimenti agli stessi operatori, ma soprattutto dando una cornice giuridica che sia nello stesso tempo rispettosa della normativa europea e che guardi a questo settore in modo particolare, eliminando gli orpelli del passato e prefigurando un'industria moderna, capace di rispondere oggi alle esigenze del settore turistico nella specificità del settore balneare, con criteri nuovi, oggettivi, che contemperino l'esigenza di realizzare un salto di qualità,

sul territorio nazionale sono circa 28.000 le strutture turistico-ricettive balneari che occupano nel periodo estivo non meno di 300.000 persone, alle quali vanno aggiunti tutti i soggetti impiegati nell'indotto,

Dobbiamo anche ricordare, a favore di chi talvolta lo dimentica, che il decreto di attuazione del cosiddetto federalismo demaniale, approvato nel maggio dello scorso anno, ha devoluto alle Regioni competenze in materia di gestione

Anche l'indagine conoscitiva diventa dunque un fatto importante, che dimostra come il Parlamento segua con grande attenzione questo settore. L'incertezza normativa ha generato un blocco degli investimenti, un blocco degli investimenti, in quanto il sistema bancario, in assenza di norme certe, non finanzia più le strutture che insistono sulle concessioni demaniali, gettando in una profonda incertezza i titolari delle stesse e determinando una drastica diminuzione del valore commerciale delle aziende. Anche questo aspetto è abbastanza preoccupante e va sottolineato.

trovare un sistema per riconoscere al concessionario, in caso di devoluzione delle opere allo Stato, un *quid* che tenga conto dell'investimento e del lavoro fatto.

tenendo conto del progresso tecnologico che caratterizza questo tipo di concessione; infine, serve un sostegno forte al Governo perché continui l'operazione che sta portando avanti il ministro Fitto con le Regioni, fermo restando che dovremmo immaginare un percorso per arrivare ad una legislazione complessiva in un quadro normativo certo, perché abbiamo quattro anni a disposizione, ma sappiamo tutti quanti che i quattro anni diventano poca cosa rispetto all'obiettivo che vogliamo perseguire.

mi rivolgo anche a tutti coloro che con un po' di patema d'animo ed un po' di preoccupazione in questo Paese ci stanno ascoltando, magari con più attenzione dei colleghi dell'Aula), il Gruppo dell'Italia dei Valori vuole approfittare di questo dibattito sulle concessioni demaniali marittime teso a chiedere al Governo impegni precisi in vista di una necessaria e non più rinviabile riforma - anche per sollevare problematiche che a nostro avviso l'Esecutivo da subito potrebbe tentare di affrontare in sede europea.

decisione di trascorrere le vacanze al mare in Italia deriva non soltanto dall'apprezzamento per la bellezza delle nostre coste, ma anche dal fatto di trovare negli stabilimenti balneari quella varietà di offerta e qualità dei servizi che rendono unici le nostre spiagge e il nostro turismo balneare. Stando ai dati della Federazione italiana imprese balneari, sul nostro territorio sono presenti circa 30.000 imprese, che vengono gestite sul demanio marittimo, fluviale e lacuale, in regime di concessione, garantendo lavoro a quasi 500.000 addetti, con 450 milioni di servizi erogati nell'arco di tempo che va da giugno a settembre: un movimento economico che si può quindi stimare intorno ai 5 miliardi di euro. Le imprese che operano sul demanio marittimo si trovano attualmente a dover affrontare, oltre all'incertezza economica per il ciclo sfavorevole, anche e soprattutto l'incertezza normativa che riguarda la loro operatività e la loro stessa sopravvivenza. Le imprese che hanno dato vita al modello italiano di balneazione attrezzata, fondamentale punto di forza della nostra competitività nel mercato internazionale per le vacanze, ad oggi restano "aggrappate" alla proroga disposta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 194 del 2009, il famoso milleproroghe. Il rischio concreto, cari colleghi, è la fine di un sistema di impresa unico ed esclusivo in Europa e nel mondo. È di tutta evidenza quale gravissimo danno si creerebbe per l'economia del Paese con la brutale "scomparsa" di 30.000 piccoli imprenditori e delle relative famiglie. In altri termini, un vero e proprio problema sociale; Noi siamo consapevoli - e lo affermiamo nella mozione - che è in corso la procedura d'infrazione notificataci dalla Commissione europea che ci chiede di conformare la nostra normativa con l'ordinamento comunitario, e in particolare con la direttiva Bolkestein. La Commissione ha ribadito che le disposizioni italiane sono palesemente contrarie alla normativa europea, in particolare su due punti: l'articolo 12 della direttiva sui servizi nel mercato interno e l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato nel territorio di un altro Stato membro. È ovvio che condividiamo la necessità di chiudere al più presto la procedura di infrazione, ma dobbiamo anche considerare che la normativa italiana negli anni ha determinato nelle imprese balneari la legittima aspettativa di avere davanti un orizzonte temporale lungo ben più lungo del 2015 - per poter effettuare gli investimenti necessari all'ammodernamento e al rinnovamento delle strutture e delle attrezzature. L'ordinamento italiano, infatti, attraverso il diritto di preferenza prima e il diritto di insistenza dopo, ha sviluppato un principio di stabilità del rapporto concessorio a cui si sono fino ad ora ispirate le stesse linea di politica economica del settore. L'attuazione di tale principio ha rappresentato una spinta alla specializzazione delle imprese del settore stesso. Da qui la necessità di costruire urgentemente, sotto forma di leggi, assieme alle Regioni e alle organizzazioni delle imprese, un nuovo sistema di regole omogenee volto a disciplinare le modalità di utilizzo del demanio marittimo lacuale e fluviale a fini turistico-ricreativi. La Commissione europea ha osservato, infatti, che la normativa italiana, oltre a violare i principi comunitari, ha creato un quadro giuridico ambiguo per gli operatori economici. la Commissione ha ricordato che, conformemente al principio della certezza del diritto, le norme giuridiche devono essere chiare, precise e prevedibili nei loro effetti. Allo stato attuale pare più che evidente, invece, che a livello sia nazionale che regionale si faccia fatica a trovare soluzioni per risolvere la problematica indicata: quindi non è una cosa semplice. Non pare infatti una soluzione decisiva la sola proroga delle concessioni al 2015; basti per questo citare il precipitato cautelare del TAR Sardegna, per il quale essa «non appare coerente con i principi comunitari in materia di trasparenza, non discriminazione e libertà di stabilimento». Tali misure necessitano, lo ribadisco, di un ulteriore intervento legislativo. A tale proposito voglio ricordare, come già detto da altri colleghi e in altre mozioni, che alla luce delle problematiche precedentemente segnalate le Commissioni riunite 8a e 10a del Senato hanno ritenuto opportuno avviare un'apposita indagine conoscitiva. L'urgenza di costruire il nuovo quadro normativo per l'intero settore era già stata segnalata nell'ottobre 2010 dalla Conferenza delle Regioni nel documento preparatorio alla IV Conferenza nazionale sul turismo; mi preme sottolineare che, nonostante gli impegni presi dal ministro Brambilla in quella sede, nel codice del turismo contenuto nello schema di decreto da poco passato al vaglio delle Commissioni nulla si dice in proposito: è come se il turismo balneare non esistesse. In sede di Conferenza sul turismo, le Regioni chiedevano un provvedimento che fosse in grado di assicurare quelle certezze di durata e di sopravvivenza che rappresentano la condizione indispensabile per favorire investimenti e crescita delle imprese interessate. L'esistenza di un rilevante settore di mercato delle concessioni di demanio marittimo e la specificità del nostro settore turistico balneare dimostrano quindi la necessità di attivarsi presso le competenti sedi istituzionali europee al fine di concordare su un impianto normativo nazionale, derogatorio, sì, a quello comunitario contenuto nella direttiva, ma comunque, colleghi e Governo, rispettoso dei principi generali dello stesso ordinamento comunitario. È quello che chiediamo nella nostra mozione. Abbiamo tempo fino al 28 dicembre 2011 per farlo: mi sembra un tempo sufficiente. Contemporaneamente, occorrerà prevedere una normativa quadro nazionale che garantisca uniformità di legislazione regionale - siamo anche in presenza del demanio regionale, del federalismo - su tutto il territorio e che fornisca criteri e modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime certi e non sovrapponibili, istituendo un tavolo di concertazione con le Regioni e i rappresentanti delle organizzazioni di settore. Noi siamo pronti a sostenervi in ogni iniziativa mirata a non penalizzare il settore turistico balneare ed i relativi livelli occupazionali e siamo disponibili, laddove ci siano le motivazioni di fondo, a cogliere la possibilità di arrivare anche a una mozione unitaria, perché il tema che è sul tappeto è importantissimo e riguarda la prima industria nazionale, cioè il turismo.